Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame affronta il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. Durante l'esame in Commissione sono state svolte numerose audizioni, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima, dato che un testo simile era stato approvato dal Senato in prima lettura nella scorsa legislatura. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che al comma 2 elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne. L'elenco delle attività vietate dal suddetto comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1, nonché alle acque salse, salmastre o lagunari.

Per le acque interne non ricomprese nell'allegato viene disposta una nuova lista di divieti, che introduce un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-*bis.* Oltre all'esercizio della pesca professionale, vengono vietati l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva e l'uso di esplosivi, elettricità e sostanze tossiche, nonché lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui può essere autorizzato l'uso di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-*quater* consente inoltre alle Regioni di autorizzare l'esercizio della pesca professionale nei laghi non inseriti nell'Allegato 1, nei quali sia già inserita la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Le altre modifiche riguardano i commi dal 3 al 7 dell'articolo 40 e mirano ad adeguare al nuovo impianto normativo quanto già previsto a legislazione vigente. In Commissione era stato approvato l'emendamento 1.10, che individuava un vincolo di destinazione per i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni commesse.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, tutelare la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali riveste un valore assoluto e significa operare direttamente per garantire benessere e salute al pianeta e a tutta la comunità umana. Questo è ancor più vero se pensiamo che proprio in Italia la biodiversità raggiunge valori elevatissimi. I nostri ecosistemi contano metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali presenti in Europa, come emerge anche da un recente *report* del WWF sulla biodiversità. Le acque interne italiane rappresentano un ecosistema ricchissimo di biodiversità, una ricchezza però che rischia di sparire velocemente. Una delle principali minacce alla biodiversità è rappresentata infatti dal bracconaggio, che è il più generale dei cosiddetti crimini di natura (*wildlife crime*). Ormai da diversi anni, tutte le acque interne del nostro territorio nazionale sono interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, finisce per essere collocato principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. In alcune province del Nord Italia, fiumi grandi e piccoli vengono ripetutamente saccheggiati da bande di predatori, pescatori di frodo, quasi tutti stranieri dell'Est Europa, che con mezzi vietati particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico, pescano di tutto e rivendono al mercato nero. Tra i mezzi più dannosi ed atti a stordire e catturare le prede, ci sono anche l'utilizzo di correnti elettriche e di bombe, come diceva prima la collega Bizzotto, di veleni e altre sostanze chimiche. si stima essere di almeno tre milioni di euro l'anno, senza contare le violazioni alle norme sanitarie, l'evasione fiscale, lo scarico abusivo di rifiuti, i furti e i danneggiamenti. Insomma, una vera e propria fiera dell'illegalità, che un Paese serio non intende più tollerare, lasciando che bracconieri e pescatori di frodo possano continuare a rovinare i nostri preziosissimi ecosistemi naturali e fluviali, orgoglio della nostra Nazione e vanto a livello mondiale per bellezza, biodiversità e varietà del patrimonio ittico. Certo, basta soffermarsi qualche istante sul valore economico che si cela dietro, per esempio, alla pesca abusiva di vongole veraci, per comprendere pienamente la portata di questo *business* illegale. Oggi un chilogrammo di vongole veraci nei punti vendita italiani può costare dai 12 ai 20 euro, ma il prezzo può variare anche in maniera considerevole a seconda della località e del periodo, potendo fruttare dai 30 ai 50 euro al chilogrammo; vongole diventate anche rarissime a causa di un predatore naturale qual è il famigerato - salito alle cronache - granchio blu. Si comprende allora perché il bracconaggio ittico non rappresenti, quindi, una semplice piaga per la filiera alimentare e per i nostri ecosistemi, ma incida in modo fortemente negativo anche su tutto l'indotto economico riconducibile al settore della pesca sportivo-ricreativa, costituito da migliaia di attività commerciali, di aziende produttrici, di strutture ricettive, operatori turistici, associazioni di volontariato, eccetera. Oltre 100.000 persone, infatti, praticano ogni anno attività agonistiche legate al settore della pesca sportiva, movimentando un giro d'affari di circa 3,4 miliardi di euro. Per questo, con il disegno di legge in discussione, che si pone in stretta continuità con il provvedimento approvato qui in Senato all'unanimità la scorsa legislatura, ma che non ha potuto vedere la luce, come sappiamo, per la sua fine anticipata, vogliamo scrivere la parola fine a reati odiosi, come appunto il bracconaggio ittico. Lo facciamo prevedendo un irrigidimento delle sanzioni in materia di bracconaggio ed un generale divieto della pesca professionale nei fiumi e nei canali italiani, consentendo però la pesca professionale in molte acque dolci, cioè in tutti quei bacini che storicamente hanno una tradizione, un indotto economico ed una filiera enogastronomica da preservare, e anche in tutte le acque salmastre e dove operano pescatori di professione, perché chi opera in maniera legale possa continuare a farlo senza alcuna intimidazione, perché, colleghi, per noi la legalità non è solo una questione di *photo opportunity*. Le disposizioni del provvedimento introducono anche una serie di divieti con violazioni che comportano sanzioni che vanno dall'arresto, da due mesi a due anni, all'ammenda

Grazie a loro, la nostra fauna e la nostra biodiversità, ma anche le nostre tavole, sono ogni giorno più sicure. Annuncio quindi che, come Gruppo Civici d'Italia-Coraggio Italia-UDC-Maie, voteremo a favore di questo provvedimento, perché si possa finalmente scrivere la parola fine al fenomeno del bracconaggio e perché i nostri rinomati e preziosi prodotti ittici, nonché tutti i professionisti del settore, possano avere una tutela in più, quella di una Stato che non arretra di fronte all'illegalità, che non cede di fronte alla violenza di chi vuole fare scempio dei nostri meravigliosi territori fluviali e lagunari.

acque interne. Si continua a parlare di pesca sportiva. Non credo che la pesca sia uno sport. Il termine pesca sportiva è un retaggio di un tempo passato in cui si interpretavano la pesca e la caccia come sport. Non è però più questo il tema. Oggi la pesca è un'attività che ha senso solo se aiuta a conservare la biodiversità. Coloro che quindi praticano la pesca nel tempo libero devono essere considerati *partner* della pubblica amministrazione per quanto riguarda il presidio

succede da un po' di tempo a questa parte, vengono aumentate, ma il problema è che non si incrementa il numero di coloro che devono controllare. Se allora non ci sono quelli che controllano, possiamo mettere le sanzioni che vogliamo, ma è complicato scovare quelli che infrangono la legge e sottoporli alla giusta sanzione. È quindi un provvedimento che pur fissando alcuni concetti assolutamente condivisibili, non va al nocciolo del problema, cioè valorizzare

a coloro che sono preposti al controllo - le Forze dell'ordine, meritevoli di tutte le nostre attenzioni e la nostra riconoscenza - le strutture e i numeri per poterlo svolgere. Il provvedimento non si preoccupa per nulla di tutto questo. Come sempre da quando arrivano provvedimenti di questo tipo dalla maggioranza, esso si limita a inasprire pene e a fissare meglio l'elenco delle cose che non si possono fare. Non posso condividere questo spirito e quindi il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

legge in discussione riprende un disegno di legge che era già stato esaminato nella passata legislatura e che, per la fine anticipata della della stessa, non ha potuto vedere la doppia lettura. Prendiamo atto e ringraziamo la maggioranza di aver preso spunto da una proposta di legge già esistente.

che accadrà nel nostro Paese. Forse dobbiamo cominciare a pensare e a trattare il nostro Paese come uno di quelli in cui l'acqua verrà meno e sempre più frequentemente, come in Spagna e Israele,

troppo piena di perdite. Paradossalmente in questa città gli acquedotti che funzionano meglio sono quelli degli antichi romani. Detto questo, il provvedimento cerca di porre l'attenzione sul patrimonio ittico delle nostre acque interne, forse anche poco conosciuto rispetto a quello marino. Ringrazio tutti i sindaci e tutti gli amministratori locali che cercano di far conoscere questo immenso patrimonio alle scolaresche, ai giovani alle giovani generazioni. Io sono stata eletta in un collegio bellissimo che include la città di Parma e in quel territorio il sindaco Nicola Cesari ha previsto l'acquario di Mezzani, che di Mezzani, che serve a far conoscere i pesci del fiume Po, perché spesso non conosciamo quelli che per tanti anni sono stati i pesci delle nostre acque interne e oggi che c'è il rischio che

che prevedrebbe dei controlli seri. Dobbiamo mettere in atto una rete che faccia questo, ma soprattutto serve una legge nazionale per coordinare tutte quelle leggi regionali che in materia sono nate e che hanno normato in maniera diversa un settore così delicato, perché sappiamo che questa è una delle materie concorrenti tra Stato e Regioni e le Regioni, dato che mancava una legge nazionale o comunque doveva essere adeguata, hanno provveduto autonomamente.

nelle Regioni e soprattutto perché, senza infingimenti, veniva dalla passata legislatura e non vedo perché, se nella passata legislatura avevamo votato positivamente, solo perché il Governo è cambiato dobbiamo cambiare il nostro giudizio. Per questo il nostro voto sarà favorevole.

Questo disegno di legge nasce dalla necessità di contrastare il bracconaggio ittico, diffuso soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale, praticato prevalentemente da organizzazioni criminali straniere. Come sappiamo, il problema si è aggravato a partire dal 2012, a seguito di politiche restrittive attuate dal Governo rumeno sulla pesca nel delta del Danubio, che ha generato l'esodo di numerosi pescatori locali verso altri Paesi europei, fra cui l'Italia, dove hanno trovato hanno trovato nel fiume Po e nella zona del delta l'ambiente naturale per svolgere la propria attività illegale, favoriti anche dalla mancanza di pene particolarmente dissuasive da parte nostra. Questa finalità lascia tuttavia intravedere un limite relativo all'approccio adottato, consistente nell'eccessiva settorialità dell'intervento, che non ha ad oggetto il bracconaggio ittico in generale, ma addirittura una specifica e peculiare tipologia di attività criminale, anche circoscritta da un punto di vista geografico. Penso che avremmo potuto fare di più, soprattutto considerando lo stato di salute dei nostri ecosistemi.

cento dei fiumi e l'80 per cento dei laghi si trovano in uno stato ecologico non buono. I dati sullo stato di conservazione delle specie non sono meno allarmanti: il 30 per cento delle specie di animali vertebrati e il 25 per cento delle specie animali marine del Mediterraneo sono a rischio di estinzione. Le zone umide sono tra gli ecosistemi più a rischio del pianeta, circa il 90 per cento delle aree umide, soprattutto, è scomparso nell'ultimo secolo in Europa, in Italia solo il 43 per cento dei fiumi raggiunge un buono stato ecologico, obiettivo fondamentale della direttiva quadro acque, mentre per i laghi la situazione è ancora peggiore, con una percentuale che crolla al 20 Una delle principali cause di questa situazione critica è da ricondurre proprio al degrado degli ambienti delle acque dolci, nonostante numerose azioni di tutela intraprese a livello europeo. In questo contesto, siamo convinti che l'approccio debba essere integrato, complessivo e severo. Dovremmo avere una strategia precisa complessiva per riportare gli ecosistemi in una situazione di benessere e di sicurezza. Nonostante ciò,

Signora Presidente, il testo all'esame dell'Assemblea non ha subìto modifiche durante l'esame in Commissione, che è stato molto approfondito e che ha visto la partecipazione e i contributi di esperti e istituzioni. Il quadro emerso è quello di un fenomeno molto grave, a cui bisogna porre un freno trovando una soluzione. Secondo i dati forniti dai carabinieri, nel quinquennio monitorato sono stati effettuati quasi 54.000 controlli, ci sono stati più di 3.000 illeciti amministrativi accertati, 197 denunciati penalmente e l'attivazione di 144 sequestri penali. Si tratta di gruppi organizzati di quattro o cinque persone che muovono fino a 40.000 euro a settimana. Poiché gli interventi e le denunce dei carabinieri, come abbiamo visto, sono molti, c'è un alto *turnover* della manovalanza, mentre diventano sempre più invadenti nei confronti della fauna e dell'ambiente i mezzi usati dagli stessi bracconieri.

Le modifiche proposte dal disegno di legge sono quindi molto puntuali e vanno a cambiare l'articolo 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne) della legge n. 154 che contiene diverse deleghe, anche in campo agricolo e agroalimentare. Si interviene sui divieti nelle acque interne, specificando che ci si riferisce alle acque lagunari, e vengono elencati gli otto laghi italiani principali e i 22 minori. Viene poi introdotto un divieto totale di pesca professionale nelle acque lacustri interne. Il testo precisa che, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati la cattura durante il periodo di riproduzione della specie, l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, quindi una serie di divieti e la disciplina dei casi in cui si può autorizzare l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività nei laghi di minori dimensioni, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Insomma, è un tema che forse a qualcuno potrebbe apparire minore, ma che ha degli aspetti fondamentali: quello di ripristinare la legalità fermando comportamenti di evidente illegalità da parte di chi si arricchisce col bracconaggio ittico; quello di tenere nella giusta considerazione l'economia di molti territori legati alla vita e all'ambiente dei laghi. Si parla quindi di legalità, di economia, di ambiente; temi che stanno a cuore a Forza Italia e al centrodestra e su cui abbiamo già lavorato e continueremo a lavorare per tutta la legislatura. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

colleghi, signor Sottosegretario, stiamo trattando un provvedimento che ha l'ambizione di debellare delle pratiche che non possono certamente essere ricondotte alla pesca, ma a veri e propri abusi su tutta la fauna ittica di fiumi, laghi e lagune, metodi di cattura invasivi e devastanti quali gli elettrostorditori, oppure veleni e fertilizzanti agricoli usati per indirizzare i pesci nelle trappole, nelle reti a tramaglio. Sembra una situazione perfetta per una scena apocalittica di un film; purtroppo, invece, sono condizioni che si ripetono e spesso nella nostra realtà. Spietati pirati delle acque utilizzano questi terribili mezzi per fare bottino nei nostri specchi d'acqua. Si utilizzano metodi brutali che ovviamente uccidono ogni essere vivente che si trova nel loro raggio di azione e che permettono, in poche ore, di avere un pescato molto consistente, con gravissime conseguenze per l'ambiente e per la biodiversità del sistema acquatico. I bracconieri, in una sola notte d'azione, riescono a fare piazza pulita di tutta la fauna ittica presente nel territorio individuato, perché dove passa l'elettrostorditore non resta nulla. Un fenomeno che, sì, è fortemente presente in molte province del Nord, ma non solo. Lo scorso dicembre è stata fatta una vera e propria mattanza lungo il fiume Tevere, nel territorio comunale di Baschi, in provincia di Terni: tre quintali di pesce catturato illecitamente proprio attraverso l'ignobile ausilio delle scariche elettriche. L'identikit dei responsabili è ormai definito: si tratta di pirati che arrivano per lo più dall'Est Europa. La ragione va ricercata nel fatto che il Danubio è finito sotto strettissima osservazione e pescare di frodo è diventato più semplice e più redditizio proprio in Italia. Così si è drammaticamente affermata, proprio negli ultimi anni, la presenza insostenibile di bracconieri nei fiumi. Questa sequela di scorribande e di saccheggiamenti ha un nome ben preciso: parliamo della piaga delle zoomafie, vale a dire lo sfruttamento e lo sfinimento delle risorse animali e quindi naturali come *business* della criminalità organizzata. Un giro che può arrivare a fruttare dai 20.000 ai 40.000 euro a settimana per ogni gruppo operativo e che rappresenta una vera e propria economia parallela parallela rispetto alle attività lecite. Si stima un affare annuale pari ad almeno tre milioni di euro; un'occasione di profitto che vanta un esercito di pescatori paramilitari pronti a tutto, perfino a usare intimidazioni e minacce verso gli addetti ai controlli. Dunque è inutile dire che il provvedimento normativo che oggi ci accingiamo a votare è stato fortemente atteso. Già nella passata legislatura ci siamo impegnati per definire un testo chiaro ed efficace, affinché non ci fossero dubbi interpretativi. Spiace constatare che il MoVimento 5 Stelle sia stato l'unico Gruppo, qui in Senato, ad aver presentato emendamenti, come se queste problematiche fossero troppo lontane da noi o ritenute di facile soluzione o, peggio, di scarsa importanza. *(Applausi)*. Davvero ritenete che questo testo sia perfetto? Sinceramente noi, fin dalla prima lettura, abbiamo ritenuto che ci fossero dei margini di miglioramento, sotto diversi profili. Uno di questi, probabilmente quello che salta maggiormente all'occhio, è quello relativo ai profili derogatori. Non si può infatti vietare una condotta e poi trovare subito l'eccezione. Parlo della deroga per la pesca delle specie eurialine, nonché per la pesca dei gamberi di fiume. In questo caso specifico il disegno di legge prevede che le Regioni e le Province autonome possano derogare al divieto di pesca professionale e al divieto di uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Il testo del disegno di legge opera poi un distinguo sanzionatorio riguardante la pesca in laghi, acque salmastre o acque interne, cioè fiumi e canali. Alcune condotte infatti sono punite con arresto e ammenda, altre invece solo con sanzione amministrativa. Il nostro intervento è stato quello di uniformare le sanzioni, prevedendo per tutte l'arresto o l'ammenda. La ragione è semplice: dare forza all'azione deterrente delle sanzioni stesse e quindi alla prevenzione degli illeciti. Prevenire è sempre meglio che curare. In questa ottica, il sequestro e la confisca di natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato devono essere disposti sempre e non solo in caso di recidiva. Un pescatore di frodo che non ha il suo barchino, infatti, difficilmente potrà continuare a fare bracconaggio. La questione andrebbe recisa sul nascere, togliendo gli strumenti funzionali a perpetrare gli illeciti. Ancora, sempre nello stesso filone, abbiamo proposto sanzioni più severe e revoca della licenza di pesca quando c'è la reiterazione delle condotte vietate, non la sola sospensione. Inoltre, per far sì che le disposizioni siano rispettate, ci deve essere anche il giusto controllo. Per questo abbiamo proposto l'estensione delle funzioni di vigilanza a tutti i soggetti istituzionali e volontari che già si occupano di vigilanza faunistica venatoria e che sono in possesso di esperienze specifiche. In questo modo viene assicurato il raggiungimento della finalità della legge, affinché le intenzioni del dettato normativo non rimangano lettera morta. Mi spiace infine per una proposta a mia prima firma approvata dalla 9a Commissione, ma che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Mi riferisco alla destinazione nell'apposito fondo antibracconaggio dei proventi derivanti dalla violazione dei divieti in materia di bracconaggio ittico. Si tratta di un fondo che esiste dal 2016 e che sarebbe stato direttamente rimpinguato dalle somme delle sanzioni irrogate. Tale proposta aveva due obiettivi sostanziali: assicurare la veicolazione sinergica delle risorse e garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e, quindi, al bracconaggio ittico nelle aree interne. Insomma, noi ce l'abbiamo messa davvero tutta per migliorare un testo che aveva bisogno di limature e l'abbiamo fatto studiando nel dettaglio le disposizioni e il punto di caduta di tali disposizioni. Al solito, i margini di ascolto sono stati pari a zero. Il nostro intervento emendativo era inoltre teso a licenziare un testo coerente anche sotto il profilo terminologico. Basti pensare che nelle righe di tale proposta si parla indifferentemente di specie ittiche, di altri organismi acquatici, di fauna ittica, e poi generalmente di animali, quando sarebbe bastato utilizzare sempre la medesima dizione, quella di fauna acquatica, per non ingenerare dubbi interpretativi. disegno di legge che si concentra sulla modifica di un solo articolo: come sappiamo, si tratta della modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, ma i cui commi si avviluppano su se stessi generando poca chiarezza e forti contraddizioni, che poi vengono formalizzate con la legge. È un disegno di legge pieno di scappatoie, come ormai queste destre ci hanno abituato. Il divieto vale per la mano sinistra e non vale per la mano destra: forse è proprio questo che guida i provvedimenti delle destre al Governo oggi. *(Applausi)*. Per tutte queste ragioni, non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto di astensione

da ormai una decina d'anni, nei fiumi e canali del Nord Italia è diffuso il fenomeno del bracconaggio ittico, cioè della pesca di frodo. Il fenomeno è diffuso in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia-Romagna e soprattutto nel Delta del Po. I bracconieri ittici provengono in larga parte dalla Romania e da altri Paesi dell'Est Europa, come Bulgaria e Moldavia. In due o tre ore riescono a pescare oltre 5-600 chilogrammi di pesce. Nelle reti finiscono carpe, pesci siluro, lucioperca, temoli russi, carassi e quant'altro, che sono destinati ai banchi dei mercati dell'Est Europa oppure - e non è raro - anche a qualche mercato italiano. Le bande di pescatori di frodo - così le dobbiamo definire - si sono spartite il territorio, non entrano mai in contrasto tra loro e hanno confini ben definiti. Ogni gruppo è composto da una decina di persone, divise in due squadre. I bracconieri arrivano sull'argine del fiume di notte e gonfiano un gommone; quindi mettono in funzione l'elettrostorditore, un congegno piuttosto semplice composto da una batteria per automobili collegata a un trasformatore regolabile. Basta immergere l'asta nell'acqua per liberare le scariche. I pesci vengono storditi e attirati verso le reti. I bracconieri in una sola notte di pesca riescono a catturare buona parte della fauna ittica presente in quell'area del fiume o del torrente. Un altro gruppo è incaricato di portare il pesce in una zona vicina, dove avviene una prima sommaria lavorazione. Poi i pesci vengono caricati in cassette colme di ghiaccio su furgoni diretti nell'Est Europa. Le norme igienico-sanitarie sono totalmente assenti. Le certificazioni per i prodotti trasportati sono spesso false. Nel Nord Italia il fenomeno è diventato importante a partire dal 2012, quando quella che in Romania viene chiamata mafia del pesce iniziò a spostarsi verso i corsi d'acqua italiani. Questo perché il Delta del Danubio, dove agivano prima i bracconieri, nel 2012 fu riconosciuto riserva della biosfera e patrimonio dell'UNESCO. I controlli aumentarono e così le pene per chi veniva trovato a pescare di frodo si sono innalzate. In Romania si rischiano oggi fino a quattro anni di carcere per il bracconaggio ittico e agiscono dodici corpi speciali impegnati nella tutela dell'ambiente. Il disegno di legge in esame interviene proprio per affrontare il fenomeno, sempre più dilagante, della pesca illegale e del bracconaggio ittico. Ma non ci sono solo questi bracconieri dei fiumi ed occorre tutelare in modo cogente la fauna ittica. Noi esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, perché è importante soprattutto l'*iter* iniziato nella scorsa legislatura. Io voglio ringraziare il senatore Simone Bossi, insieme al collega Campari,

per l'attivismo, e soprattutto gli uffici legislativi e tutti i colleghi in Commissione, perché siamo riusciti, in tempi brevissimi, a chiudere il cerchio su una problematica molto importante. Sul testo sono state svolte numerosissime audizioni da parte della Commissione, dalle quali è emersa la necessità di intervenire quanto prima per ripristinare lo stato di legalità, attraverso l'introduzione di semplici ma specifiche norme relative ai controlli per la salvaguardia del patrimonio ittico e al contrasto al bracconaggio. Il disegno di legge si compone di un unico articolo, di modifica dell'attuale articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il cosiddetto collegato agricoltura, intende porre fine a tale situazione. L'articolo 40, come modificato dal presente disegno di legge, elenca le attività vietate nelle acque interne. Con le modifiche proposte viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne: questo diventa fondamentale.

Per le acque interne non ricomprese in tale allegato viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti. In particolare, oltre all'esercizio della pesca professionale e all'uso dei relativi strumenti e attrezzi, viene vietato l'uso e la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relativo alla specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. In ogni caso - come è stato detto bene in precedenza - non è un limite aver dato la possibilità, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle Regioni autonome, di intervenire per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o comunque tradizionale. Si tratta, dunque, di un disegno di legge di buon senso, condiviso sia dal mondo della pesca sportiva che dal mondo della pesca professionale, che chiedono regole certe e più stringenti nell'esercizio dell'attività di pesca. Un ringraziamento va a tutte le guardie volontarie, che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro presenza, rischiando in alcuni casi la vita di fronte a bande armate di bracconieri, senza la possibilità, con le leggi vigenti, di poterle fermare. Ringraziamo il corpo dei carabinieri forestali, che hanno gestito in modo attento le operazioni di vigilanza, in collaborazione con la vigilanza FIPSAS. Grazie alla Federazione italiana pesca sportiva e al presidente Matteoli, hanno messo a disposizione tutte le risorse per contrastare in ogni modo questa ripetuta mattanza, che si ripete ancora - badate bene - ogni notte sulle nostre acque. In questi anni c'è stato un grande lavoro di cooperazione tra tutte le parti, che ha permesso di effettuare operazioni importanti di salvaguardia della fauna ittica. E guardate che il tema della biodiversità si collega anche a questo, perché il mantenimento della fauna ittica e l'applicazione di norme razionali

Vorrei iniziare dalla parte finale dell'intervento del senatore Bergesio. È indubbio e indiscusso che i fenomeni di abusivismo e di bracconaggio

delle acque disponibili. È pertanto più facile per i fenomeni criminosi poter intervenire e creare danni irreparabili alla nostra biodiversità.

quello ittico ma in tutti i campi. Pensiamo alla vespa velutina, che sta falcidiando i nostri alveari, al punteruolo rosso, al cinipide del castagno e a tanti altri parassiti che arrivano nei nostri territori e distruggono un patrimonio essenziale dal punto di vista produttivo e di biodiversità del nostro ambiente.

Il provvedimento in esame, come esposto, serve anche per combattere gravi fenomeni criminali. È su questo che io vorrei puntare, insieme al fatto che è un provvedimento anche di tutela igienico-sanitaria. Noi ci dobbiamo interrogare se due fenomeni contingenti e urgenti, come la tutela igienico-sanitaria del consumatore rispetto a un prodotto la cui certezza nella filiera di trasformazione non è garantita e le scorribande di criminali,

prevedere delle mere sanzioni amministrative per talune fattispecie è di per sé insufficiente. Credo che, rispetto ai comportamenti, ci sarebbero dovuti essere una graduazione diversa delle pene, anche per l'ipotesi della recidiva, e l'individuazione di delitti. Siamo infatti in presenza di vere azioni criminali. E non lo dico

Un plauso va sicuramente a tutto il mondo del volontariato, alle guardie volontarie, agli organismi delle varie associazioni della pesca e quant'altro. Ma è certo che, di fronte a fenomeni criminali di bande specializzate, che operano in campo aperto, spesso in orari notturni, noi non possiamo rimetterci solo alla buona volontà di volontari. Si tratta di soggetti organizzati e il contrasto a questo

Sul tema delle Province, troppo spesso concentriamo l'attenzione sugli organismi politici, ma il vero tema sono gli organismi tecnici la necessità di dare risorse all'ente Provincia affinché possa implementare la dotazione del proprio personale e fare quello che è uno dei suoi compiti istituzionali, ossia il controllo in campo aperto sia in ambito faunistico-venatorio, sia in campo ittico e quant'altro.

alle risorse affinché i controlli possano essere eseguiti. In caso contrario, rischiamo di avere un provvedimento che nel merito

il disegno di legge di modifica dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 pone un punto importante nella lotta al bracconaggio ittico.

con paesi italiani e diede avvio a questo fenomeno che risale a più di dieci anni fa, pur essendo la legge del 2016.

Bergesio. Iniziative di carattere sanzionatorio, ma che sono per lo più di carattere amministrativo, non sono sufficienti. Non possiamo pensare che siano sufficienti. Va bene fare questo passaggio, ma è inevitabile poi arrivare all'aspetto di carattere penale della questione. Si diceva che in Romania si arriva fino a quattro anni di reclusione. Oggi che cosa avviene? Si aumentano le sanzioni e si arriva al sequestro del mezzo

Signor Presidente, per arrivare alla conclusione del mio intervento, ritengo questo un passaggio fondamentale, ma prodromico ad un altro, perché sarebbe come dire

ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile

elezioni e delle immunità parlamentari, a maggioranza, ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto

copia degli atti del procedimento civile numero registro generale 32914/2021, pendente nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se le condotte oggetto del procedimento civile *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento. Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta il 18 ottobre 2023 e l'ha annunciata in Aula in pari data. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 14 novembre e del 13 dicembre 2023, nonché del 16 e del 23 gennaio gennaio 2024, deliberando in tale data nel senso della insindacabilità. Sul fatto, signor Presidente, la vicenda *de quo* è già stata sottoposta all'attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura e, in data 26 ottobre 2021, la Giunta, in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli, ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nel corso della seduta d'Aula del 16 febbraio 2022 fu accolta la proposta di rinvio dell'esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite. Avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento, l'ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse *ex* articolo 68. Il tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato Nella seduta di Giunta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha ritenuto di condividere le conclusioni della relazione per l'Assemblea, depositate nella scorsa legislatura dal senatore incaricato Pellegrini, nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, della garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68. Nella seduta del 13 dicembre 2023, alla luce del dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta, la relatrice ha dichiarato di rinunciare all'incarico. preso avvio da un *post* pubblicato su Facebook in data 7 dicembre 2018, con cui l'allora senatore Lanzi criticò la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare nel dicembre 2018 il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle per aderire al Gruppo dei dei deputati di Forza Italia. L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dileggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a lui causato. L'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il bersaglio da delegittimare ai fini di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica. politica. Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre inscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione, introducendo introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientravano quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del regolamento interno al Gruppo. Ha richiamato, peraltro, le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare, tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del consiglio direttivo direttivo dell'8 ottobre 2018. Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza. In particolare, in quanto membro del direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle, le espressioni da lui utilizzate, le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole

Colleghi, siccome siamo chiamati a votare e tra l'altro, conoscendo il contenuto della relazione, il passaggio che sta illustrando il collega Sallemi è particolarmente importante, anche frutto di una discussione con qualche apporto di novità, vi chiederei di prestare attenzione. Prego, senatore Sallemi, e mi scusi per l'interruzione. SALLEMI, *relatore*. Grazie, Presidente. Come dicevo, costituiva, ad avviso del richiedente, manifestazione *extra moenia* del proprio pensiero politico già espresso in precedenza nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Secondo il giudice del caso di specie, il piano di attività del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento. Pertanto, ad avviso dell'autorità giudiziaria, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate a una sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad un'attività politica del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. In punto di diritto, Presidente, la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* - ad esempio un'intervista - da un parlamentare siano coperte dalle prerogative dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito dell'attività parlamentare. In altri termini, la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgative di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del consiglio direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Gruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano, ma passavano ad altro Gruppo. Il senatore chiese a tal proposito che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato. La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita - citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso - nel corso della riunione del consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018. Tanto premesso, sono condivisibili, in riferimento al caso in esame, le conclusioni contenute nella relazione predisposta dal senatore Paroli nella scorsa legislatura, che fu illustrata dal presidente Gasparri nella seduta della Giunta svoltasi il 26 ottobre 2021. In tale sede è stato opportunamente precisato che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura bivalente, essendo associazioni privatistiche, ma svolgendo al contempo funzioni squisitamente parlamentari e quindi pubbliche per eccellenza. Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* e atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere conseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso. Nel caso di specie il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del consiglio direttivo del Gruppo dei senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta peraltro essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su Facebook che porta la data del 7 dicembre 2018. In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti alternativi tra loro, ossia preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare sulla base delle specifiche situazioni. Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità delle prerogative dell'insindacabilità del caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel consiglio direttivo del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018. Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

il Gruppo MoVimento 5 Stelle dissente dalle conclusioni del lavoro istruttorio svolto dalla Giunta e dalla relazione del relatore. Appare evidente che, pur trattandosi di un parlamentare del nostro Gruppo, non avremo atteggiamenti ondivaghi. Noi esaminiamo ogni singolo caso e giungiamo alle nostre considerazioni non in virtù di meri convincimenti personali o su ragionamenti basati sull'opportunità politica del momento; bensì ci atteniamo - e ci atterremo anche in questo caso - a consolidati orientamenti degli organi che plasmano la giurisprudenza dell'attività della Giunta. Sarebbe pleonastico entrare nel dettaglio e illustrare le ragioni del nostro convincimento e il motivo è presto detto. Se ci trovassimo di fronte ad un organo effettivamente paragiurisdizionale, avremmo in tutte le sedi mosso dei convincimenti tecnici che avrebbero potuto far emergere un indirizzo interpretativo che avrebbe consentito all'ex senatore Lanzi di far valere, in sede processuale, la scriminante dell'esercizio del diritto, nello specifico l'esercizio del diritto di critica politica, in tal modo escludendo la configurabilità stessa del reato. Le conclusioni delineate dalla Giunta creano un vasto ambito inesplorato, il quale dovrà essere colmato proprio da coloro i quali stanno innovando così profondamente la prassi e questo, obiettivamente, mi preoccupa e non poco. Mi spiego. La Giunta ha interpretato in senso assolutamente estensivo la pronuncia della Consulta n. 2982 del 2004. La richiamata decisione, assunta come precedente volto a giustificare la presente deliberazione, attiene ad un piano logico-giuridico totalmente difforme da quello preso in considerazione dalla relazione che stiamo per votare. Infatti, in quel caso la *ratio* della pronuncia di insindacabilità per le opinioni espresse era rinvenibile nell'equiparazione della Commissione parlamentare d'inchiesta quale, nel caso di specie, la Commissione antimafia, ad articolazioni del Parlamento, in quanto parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno e con riguardo al loro funzionamento. È evidente che appare assolutamente improprio equiparare il lavoro delle Commissioni parlamentari d'inchiesta organi tra l'altro deliberati con disposizione legislativo di rango primario - a quanto avviene all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, i quali andrebbero considerati come i luoghi politici per eccellenza in cui maturano ragionamenti politici che, solo in un secondo momento, prenderanno la forma di attività parlamentare. Infatti, a differenza di quanto illustrato per le Commissioni d'inchiesta, la citata sentenza, richiamata per giunta nella relazione, è molto chiara nel definire i Gruppi parlamentari come organi politici e non parlamentari in quanto - cito testualmente - «comunque «comunque infatti si vogliano definire i Gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscono uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte

Invece, con la presente deliberazione della Giunta - e questo costituisce il precedente al quale facevo riferimento - si è teso a stabilire che siano da considerarsi atti idonei a scriminare le dichiarazioni all'esterno anche le affermazioni rese all'interno delle riunioni dei Gruppi parlamentari, qualora le stesse siano sufficientemente documentate. Ciò che importa, o meglio che dovrebbe importare ai fini dell'avverarsi della prerogativa della insindacabilità, è l'esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa e attività non genericamente politica, bensì parlamentare, parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultimo e di conseguenza quello dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definiti in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. Occorre quindi un'analisi caso per caso. Presidente, mi permetta una valutazione in generale sull'attività della Giunta, perché, seppur apprezzando la conduzione dei lavori da parte della Presidenza, purtroppo stiamo assistendo ad una prassi (si vedano gli ultimi casi trattati di Gasparri, Giovanardi, Giarrusso e Clini su tutti) che sembra rivolta alla creazione di precedenti tali da far ricomprendere qualsivoglia opinione espressa da un parlamentare all'interno della previsione dell'articolo 68, Costituzione, con l'evidente rischio di creare sacche di immunità e una sorta di privilegio di funzione, confliggendo in modo irrimediabile con i principi costituzionali fondamentali e i diritti di altri soggetti. Abbiamo affrontato precedenti assolutamente differenti, tutti però accomunati dalla medesima conclusione: la sussistenza della insindacabilità. Io mi chiedo, signora Presidente, se siamo proprio sicuri che nelle nostre decisioni non ci sia nulla da recriminare. Siamo proprio sicuri che le nostre deliberazioni siano ineccepibili? Siamo proprio convinti del fatto che non sia, all'avverarsi di determinate condizioni, una soluzione preferibile quella di difendersi in un processo e di far valere in quella Noi siamo sicuri che l'ex senatore Lanzi ben potrà far valere i propri convincimenti ed essere scriminato in virtù del riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica politica. Voi ne siete altrettanto sicuri in relazione ai vostri parlamentari? vostri parlamentari? Penso che l'attività decisoria della Giunta dovrà, auspicabilmente nel breve periodo, riallinearsi a quanto delineato dall'articolo 19 del Regolamento del Senato, dalle ultime pronunce sta emergendo un consolidato indirizzo che appare assolutamente estensivo delle prerogative parlamentari, anche in ragione della strumentalizzazione che si sta facendo del mutato esprimersi del mandato parlamentare, volto a far ricomprendere nel terreno della insindacabilità tutte le occasioni in cui il parlamentare in ogni modo raggiunga il cittadino, frustando la *ratio* originaria dell'istituto in parola e piegando le ragioni parlamentari a meri interessi politici. Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla proposta della Giunta di diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere. *(Applausi)*.

venga applicata la guarentigia dell'insindacabilità, è necessario che vi sia nesso funzionale fra le espressioni che vengono usate *extra moenia* e l'esercizio del mandato parlamentare, pur non essendoci la necessità di una corrispondenza totale, ma sostanziale.

una tendenza ad ampliare l'applicazione della guarentigia dell'insindacabilità, tenendo conto anche della modifica dei *mores* e dei modi di espressione nella politica. Questo senza voler ammettere, riconoscere, tollerare che vi siano pesanti espressioni, auspicando invece che il nostro linguaggio sia il più possibile rispettoso in un clima sereno. È chiaro, però, che il modo stesso con cui vengono rappresentati i pensieri nella nostra società deve tenere anche conto di questi cambiamenti e la Giunta ne ha preso atto.

Sorge però un problema, di cui dobbiamo prendere atto e che dovremo anche elaborare nelle sedi adatte, in particolare nella Giunta per il Regolamento.

Lanzi. Sappiamo bene come la politica si stia esprimendo e come spesso ci si esprima su questi diabolici strumenti che sono i cosiddetti *social*.

dispiaciuto per la sua salute, che è un fardello molto pesante da portarsi dietro. Questa ironia pesante sulle condizioni dell'onorevole Dall'Osso riteniamo che non possa essere considerata una critica politica; essa è anzi un'espressione abbastanza odiosa, che manca di rispetto a quelle che sono le caratteristiche e le condizioni di una persona con disabilità.

Signora Presidente, ha ragione la collega Lopreiato quando mette in evidenza che

Il caso di specie, che riguarda il senatore Lanzi, è un caso particolarmente delicato e importante, perché

che si riuniscono ovviamente in questi Palazzi. È noto che la Corte di cassazione ha riconosciuto che i Gruppi parlamentari hanno una natura ambivalente. Ci sono cioè due piani di attività dei Gruppi, uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i Gruppi parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni, e uno invece di natura politica, per cui sono assimilabili ai partiti politici. Premetto che non possiamo entrare troppo nel merito delle opinioni espresse dai singoli parlamentari, ma che dobbiamo semplicemente valutare se le opinioni espresse *extra moenia*, cioè fuori da questi Palazzi, siano state precedute, quindi in qualche modo giustificate, da interventi e atti tipici svolti in queste sedi. A meno che non si tratti di espressioni palesemente

pronunciò delle critiche, che risultano dai verbali del Gruppo parlamentare di cui allora faceva parte,

in due circostanze diverse, due riunioni diverse, il senatore Lanzi chiese che si applicassero anche le sanzioni previste dal Regolamento e dagli statuti

opinioni differenti. In questo caso, per l'esistenza di un verbale che attesta le cose che sono state dette all'interno del Gruppo; per la circostanza che si è trattato di opinioni espresse in riferimento alla composizione del Gruppo parlamentare, quindi in relazione a una condizione che attiene alla funzionalità del Gruppo parlamentare, alla sua funzione tipica e alla sua consistenza all'interno delle Aule parlamentari, riteniamo che si possa introdurre un principio che ci pare coerente anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale: quando quelle opinioni vengono espresse e sono debitamente documentate all'interno di riunioni di Gruppi parlamentari dentro questi Palazzi; quando si tratta di opinioni che vengono espresse non tanto su questioni di natura politica generale, ma su questioni che attengono esattamente alla funzione del Gruppo parlamentare, pensiamo che in questo caso sia corretto ritenere che possano ritenersi scriminate le stesse opinioni che poi vengono espresse anche fuori successivamente. Questo è il caso di specie quindi riteniamo condivisibile, sia pur riconoscendo che si tratti di materia largamente opinabile, la conclusione che ha esposto il relatore. Pertanto, voteremo a favore.

le dichiarazioni rese dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

Allegato B).* Come concordato, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo. La seduta è sospesa.

ma è una cosa a cui tenevo. Alla Conferenza dei Capigruppo, appena

la Pasqua non si celebrava a mezzanotte, ma alle ore 11 o comunque nella tarda mattinata: le campane suonavano

occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. *(Applausi)*. Questo è l'augurio che penso sia giusto rivolgere a tutti voi e più vastamente del Senato. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito il nuovo calendario dei lavori fino al 24 aprile. La settimana dal 2 al 5 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Il calendario della settimana dal 9 all'11 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione; dalla sede redigente, disegno di legge sulle disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative, approvato dalla Camera dei deputati; deputati; disegno di legge su disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di venerdì 5 aprile; aprile; dalla sede redigente, istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati. Il calendario della settimana dal 16 al 18 aprile prevede la discussione dei seguenti argomenti: disegno di legge in materia di valutazione del comportamento degli studenti, i cui emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 aprile; discussione della risoluzione approvata dalla 3ª Commissione sulla situazione politica in Venezuela, in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Nella settimana

su ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e, ove presentato in tempo utile, il Documento di economia e finanza